L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Prego, senatore Ieri, signora Presidente, il senatore Zanda ha formulato a nome del nostro Gruppo una forte ed argomentata denuncia sullo scadimento generale del procedimento e della qualità legislativa che abbiamo registrato in questi mesi e di cui questo testo costituisce un emblema, essendosi vieppiù, in sede di esame presso le Commissioni di merito, rigonfiato di norme estranee al suo oggetto, frettolosamente e reiteratamente introdotte dal relatore e dal Governo fino a qualche ora fa: ben oltre, quindi, i termini fissati per la presentazione dei testi in Commissione. noto a lei e a tutti noi, stiamo esaminando un disegno di legge collegato alla finanziaria. La disciplina del regime di ammissibilità degli emendamenti per i disegni di legge collegati alla finanziaria è dettata

il quale prevede la preventiva declaratoria di accertamento del contenuto dei disegni di legge collegati

quale prescrive l'inammissibilità degli emendamenti, di iniziativa sia parlamentare che governativa, che rechino disposizioni estranee all'oggetto di di questo tipo di disegno di legge. Tale estraneità è da valutare, lo ripeto, rispetto alla legislazione vigente nonché al DPEF e alla relativa risoluzione parlamentare. per questo tipo di disegno di legge è necessario un doppio vaglio preliminare, affidato al Presidente del Senato: quello del collegamento e quello Sottolineo che l'esame è doppio perché è evidente che, se prevalesse (com'è avvenuto e sta avvenendo, ed è questo l'oggetto del richiamo e della denuncia)

risulterebbe sostanzialmente svuotata. La *ratio* di questa norma regolamentare, di questo regime speciale è facile da individuare: i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica beneficiano di una

che dettano appunto il regime restrittivo di ammissibilità degli emendamenti, a noi risultano palesemente violate per molti aspetti e su molti

Mi limito quindi a richiamare la sua attenzione su questa necessità di esame accurato e preventivo sia in ragione della estraneità all'oggetto del disegno di legge il titolo del disegno di legge costituisce un perimetro molto ampio di materie: sviluppo economico, semplificazione, competitività, processo civile), sia relativamente a materie fatte oggetto di emendamenti che sono estranee al contenuto della risoluzione di approvazione al DPEF. Sottolineo questo aspetto, signora Presidente, perché vengono vengono introdotti temi e testi che nulla hanno a che fare con gli argomenti elencati nella risoluzione stessa. Si pone poi un problema ulteriore. Se per i testi che non sono stati approvati dalle Commissioni di merito, penso che lei, signora Presidente, non avrà alcuna difficoltà ad effettuare il problema si pone invece relativamente agli emendamenti che già sono stati approvati dalle Commissioni di merito. Questo argomento fu già affrontato, signora Presidente, nella seduta del 19 novembre 2008, allorquando noi sollevammo una questione analoga relativamente al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge.

Nel sottolineare l'esigenza di un'applicazione rigorosa della norma regolamentare relativamente al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, disse che non se la sentiva di dichiarare inammissibili emendamenti già approvati dalle Commissioni di merito, perché questo avrebbe significato un'applicazione sostanzialmente retroattiva di questo orientamento più rigoroso.

«esprimo qui (...) una forte raccomandazione ai Presidenti delle Commissioni in ordine ad un puntuale vaglio di ammissibilità degli emendamenti a decreti-legge» - la regola quindi è la stessa, signora Presidente, anche testualmente è la stessa norma regolamentare - «anche sotto il profilo richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale (...). La Presidenza si riserva fin d'ora di valutare tali emendamenti con l'opportuno rigore» - disse il Presidente del Senato tre mesi fa - «e di dichiararne se del caso l'improponibilità qualunque sia la loro provenienza, dunque anche se approvati in Commissione o proposti dal Governo». Quindi è stata assunta una decisione sul punto. Concludo, signora Presidente,

durante l'esame del provvedimento; si vuole riformare con una delega il processo amministrativo, ma non c'è traccia di questo tema nella risoluzione di approvazione del si vuole riformare il processo contabile relativamente alla materia pensionistica, quello davanti alla Corte dei conti; si vuole riformare l'Avvocatura dello Stato; si vogliono dettare norme sulla dirigenza pubblica, sulla vigilanza sui servizi sui servizi pubblici locali, sulle farmacie, sull'ENIT, sugli enti di ricerca, sui precari della Croce rossa, sulla fondazione «Ugo Bordoni», e potrei continuare ancora. mi sembra che occorra un intervento serio, risolutore, che chiediamo venga effettuato prima dell'inizio dell'esame degli emendamenti, altrimenti ci riserviamo di sollevare, volta per volta, in rapporto ai singoli emendamenti,

di aver fatto una legge finanziaria snella e quindi di non aver consentito l'introduzione di un numero elevato ed eterogeneo di norme. In realtà si susseguono provvedimenti,

bisogna osservare che il disegno di legge collegato in esame, così come trasmesso dalla Camera dei deputati e a seguito delle modifiche introdotte in sede referente dalle Commissioni riunite, costituisce riunite, costituisce un provvedimento estremamente complesso ed eterogeneo, che investe le competenze di diversi Ministeri e rende quindi non facile l'applicazione del comma 2*‑ter* dell'articolo 126*‑bis*. Tuttavia, la Presidenza, pur in presenza di un sistema normativo difficilmente riconducibile ad unità per i suoi contenuti e le sue finalità, sta valutando la proponibilità dei numerosi emendamenti presentati, dovendo tenere in ogni caso presente l'articolo 126*‑bis*, comma 2*‑quinques*, del Regolamento, che consente la ripresentazione degli emendamenti respinti in sede di Commissione. Resta comunque fermo il principio, di cui al comma 2*‑ter* del richiamato articolo 126*‑bis*, dell'inammissibilità degli emendamenti ed eventualmente di parti di testo sui quali la 5a Commissione permanente

Presidente, non commento le considerazioni del collega Ferrara perché si commentano da sole, visto che lui stesso sta ammettendo che si sta operando nel modo che denunciavo poc'anzi. Intervengo solo per

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.700, 12-*bis*.700 (limitatamente al secondo periodo), 22.700, 22.701, 23-*bis*.0.700 (limitatamente alla lettera *a)* punto 2), 26.0.700 (testo 2). Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 12-*bis*.0.700, con l'osservazione che costituisce un utilizzo improprio il ricorso alle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dalla copertura finanziaria della proposta emendativa. Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sulle proposte 9.200, 9.30, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.9, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.300 (testo 2), 19.0.400. Esprime altresì un parere non ostativo sulle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l'ultimo periodo; che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l'ultimo periodo. Esprime sulla proposta 26.0.8000 parere non ostativo con la seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre sostituire il riferimento all'articolo 3,

nonché all'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte fino all'articolo 26, ad eccezione che sugli emendamenti 19.400,

Signora Presidente, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 vogliono sottolineare l'importanza degli investimenti in banda larga per il rilancio produttivo del nostro Paese. In tutto il mondo si guarda alle nuove tecnologie della comunicazione proprio come un grande impulso per la ripresa del sistema economico. A noi pare che il Governo faccia poco in questa direzione: di qui la necessità di istituire un apposito fondo di sostegno alla diffusione della banda larga nelle aree in *digital* *divide*, che sono molto numerose nel nostro Paese, non solo al Sud ma anche al Centro e al Nord, ricordando che l'Italia è molto al di sotto europea per gli accessi in banda larga.

Il senatore Legnini ha lamentato l'eterogeneità del contenuto di questo provvedimento e, per certi aspetti, un certo grado di eterogeneità esiste;

Grazie,

di far togliere le schede laddove non c'è un senatore seduto, altrimenti per ogni votazione chiederemo la verifica. Da questa postazione si osservano quattro o cinque schede inserite, basta guardare, e mi dispiace che i senatori Segretari non se ne accorgano. alla quinta fila ce ne sono due. La prego quindi di dare questa disposizione.

**Il Senato non approva.**

Grazie, senatore Quagliariello.

Ho letto quest'estate su «La Stampa» una lettera di giovani alunni di una scuola media superiore di Torino. sarà adottato questo sistema, non invitiamo più le scuole ad assistere alle nostre sedute, perché è una vergogna che non possiamo più accettare.

Senatrice Incostante, per cortesia, ci sono i colleghi senatori Segretari preposti a questo lavoro. Andiamo avanti con la votazione.

Signora Presidente, accetto volentieri la modifica proposta dal relatore e ringrazio il Governo per il suo parere conforme

comunitaria sui servizi finanziari. Rischiavamo di stroncare quasi sul nascere il percorso, spesso svolto da giovani, di consulenti finanziari indipendenti e liberi dal conflitto d'interesse con le banche. In questo modo riapriamo la strada alla crescita di una professione che dovrà aiutare il nostro Paese, per la propria parte, ad affrontare meglio e con maggiore consapevolezza l'attuale crisi finanziaria.

emendamenti in esame è di eccezionale interesse per il mondo delle imprese artigiane, che si vedono potenzialmente tagliate fuori da una grande quantità di lavori.

il Governo è d'accordo con il relatore, tenendo presente che l'esclusione di carattere oggettivo dell'emendamento 12.0.3 trova una ragione nella limitatezza dei lavori e, quindi, nella

Una particolare tutela per questo tipo di consorzio è prevista dalla legge quadro per l'artigianato. Quindi non facciamo nulla che alteri il sistema di concorrenza con altre tipologie di consorzio di imprese.

con lo *Small business act*, che peraltro abbiamo adottato, è assolutamente coerente con le forme di aiuti che si intendono dare in modo *bipartisan* al sistema di imprese, che adesso sta pagando un prezzo più rilevante alla crisi.

innanzitutto che si sia aperto questo confronto sul tema della partecipazione delle imprese artigiane, perché è molto utile che il mondo artigiano sappia che abbiamo ben presente questi ordini di problemi e che ce ne stiamo occupando, anche con spirito costruttivo tra Governo e settori del Parlamento. Dal punto di vista dell'approfondimento, capisco che adesso, sul tamburo, varare una norma potrebbe prestarsi a qualche equivoco. Non lo nascondo e lo riconosco.

la dimensione identitaria dell'impresa (cioè quella artigiana, secondo la legge 8 agosto 1985, n. 443), con la prevalenza dell'impresa artigiana nei consorzi genericamente intesi e non specificamente artigiani, e la dimensione del *business* a cui possono

Uffici, all'ordine del giorno firmato dal collega Mugnai e da me si aggiunge ben gradita la firma del senatore Sangalli con l'integrazione che egli propone e che per parte nostra condividiamo.

possa essere contenuta anche nei Regolamenti parlamentari, in modo che possa indirizzarsi al legislatore primario, cioè al Parlamento.

meglio questo testo, magari riesaminandolo nella sede più propria, che credo sia al termine dell'esame degli emendamenti del provvedimento in

le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate, se non in modo esplicito, con l'emendamento 3.3 intendiamo suggerire il modo per essere espliciti. Indichiamo

o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga o rimanda ad altre disposizioni legislative». Se uno si limita a dire che bisogna essere chiari, ma non dice poi

3.3, testé illustrato dal senatore Pardi,

Governo,

La *ratio* è unica ed è quella di garantire, nel meccanismo della decisione, una maggiore collegialità, che invece non si coglie nel testo che tende a restringere i centri di decisione.

Signor Presidente, penso che sia sfuggito a molti colleghi, se hanno guardato solo il testo originale e non quello uscito dalle Commissioni, 5.500, che è stato approvato dalle Commissioni e quindi ormai fa parte del nostro testo. Cosa si diceva in esso? Si parlava del termine per la procedura cui hanno diritto i cittadini per una risposta, prevedendo che debba essere di 30 giorni, che per leggi di particolare complessità si possa arrivare anche a 180 giorni e poi si concludeva dicendo i termini ivi previsti non possono comunque superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. Allora, ho chiesto spiegazioni alle Commissioni, ma non mi è stata data risposta.

invece, tutti i cittadini italiani hanno diritto ad avere certezza dei tempi nei procedimenti amministrativi, tranne gli stranieri. Questi, per fare un esempio, se hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno nel novembre 2007, sono ancora lì che aspettano e non sanno quando l'avranno. Trovo che questa norma - a meno che qualcuno del Governo mi spieghi che ho capito male male - sia indegna: quindi, voteremo contro anche per questo, oltre che per tutte le osservazioni che aveva fatto precedentemente la collega Incostante.

questo emendamento, a mio giudizio, presenta spunti di grandissimo interesse: anziché ritirarlo, chiederemmo al relatore ed al Governo di valutare l'ipotesi di accantonarlo.

Colleghi, sono certo di esprimere i sentimenti dell'Assemblea nel rivolgere un pensiero di umana solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e alla sua famiglia, colpiti questa notte dall'improvvisa perdita della loro congiunta, signora Maria Antonietta.

correttivi di cautela a proposito delle dichiarazioni di inizio attività che in edilizia stanno diventando il grimaldello per costruzioni edilizie di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, in qualsiasi luogo, spesso in deroga ad una quantità infinita di provvedimenti reali. Cito, a solo titolo di esempio, quello che è successo con il caso del cinema multiplex a Firenze nella zona di Novoli, ex FIAT, dove con una sola dichiarazione di inizio attività corredata di un solo schizzo senza nemmeno un minimo di accenno di piano particolareggiato, si è costruito un palazzo di otto piani che doveva contenere da sette a otto cinema. Dato che questo è un sintomo, diciamo così, di un modo di procedere totalmente fuori dai principi, si propone di aggiungere alla fine del comma 3, dove si parla dell'inizio attività, la formula cautelare: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e al decreto‑legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni». L'intenzione è quella di garantire di garantire una corretta applicazione della legge.

un invito al ritiro

dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 5, che stabilisce che restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di

perché l'organizzazione dei servizi sanitari è competenza esclusiva delle Regioni.

per una questione che attiene anche allo stile delle norme che variamo, sarebbe opportuno eliminare questi due commi, la previsione legislativa potrebbe risultare non applicabile in ragione di atti amministrativi che le Regioni potrebbero determinare con i piani sanitari regionali. In aggiunta alla soppressione dei commi 1 e 2, chiediamo con il successivo emendamento 9.11 quanto meno la soppressione della lettera che anche in questo caso reca una previsione invasiva delle competenze regionali, in relazione alla qualificazione di ruralità delle farmacie. Tale norma è in contraddizione con l'intero articolo, perché vorrebbe sottrarre alle Regioni il riconoscimento delle peculiarità presenti nei rispettivi territori, da limitare l'azione tesa a garantire la presenza dei presidi farmaceutici sostenuti da provvedimenti regionali anche nelle realtà rurali.

una localizzazione o regionalizzazione eccessiva che, secondo noi, potrebbe addirittura avere dei profili di incostituzionalità.

la possibilità che venga estesa l'attività della farmacia intesa come presidio sociosanitario del territorio, secondo le previsioni ben definite nei punti da *a)* ad *f)*. Tale emendamento tende a rimuovere una norma del Testo

giusto obiettivo di evitare condizioni di conflitto. Stiamo parlando del 1934, epoca in cui le professioni sanitarie erano quelle del medico, del farmacista e del veterinario. Oggi le professioni sanitarie sono oltre 25.

sanitarie, consente di mantenere impregiudicato il principio dell'incompatibilità dell'esercizio delle due professioni in farmacia, quella del medico e quella del farmacista. farmacista. Resta impregiudicato cioè il principio che non è possibile che all'interno della farmacia si svolga un'attività da parte di un operatore della sanità che ha la cosiddetta legittimazione alla prescrizione, per evidenti motivi di conflitto, ma questo principio viene limitato esclusivamente a quelle professioni sanitarie che hanno la legittimazione alla prescrizione e non ad altre. Ciòconsentirebbe, per esempio, ad un infermiere di recarsi periodicamente, in orari prestabiliti, in una farmacia e

Porto questo esempio, ma potremmo portarne tantissimi altri che vanno nella direzione di consolidare la farmacia quale presidio sociosanitario del territorio. Si tratta di un ammodernamento che sembra che sembra sia condiviso in modo congiunto, che è assolutamente attuale con i tempi, che restituisce il valore e la dignità alla farmacia e la integra in modo più pieno nell'ambito dei servizi sanitari e sociosanitario-assistenziali del territorio, nel rispetto delle prerogative di carattere generale che attengono alla competenza legislativa dello Stato e della potestà legislativa in termini concorrenti delle Regioni, così come opportunamente precisato in premessa all'articolo 9. Presidente, chiedo che l'emendamento in esame possa essere considerato con la necessaria attenzione e con favore, perché va nella direzione di qualificare i servizi sociosanitario-assistenziali del territorio.

il parere è sostanzialmente conforme al relatore con una avvertenza di carattere generale. Come mi sono permesso di dire all'inizio, è vero che il è vero che il provvedimento contiene norme eterogenee. Però, questo non consente a mio sommesso avviso di rendere l'eterogeneità l'elemento caratterizzante di questo provvedimento. Nell'articolo 9 sono stati proposti emendamenti che riguardano la materia sanitaria, segnatamente l'emendamento 9.17, primo firmatario il senatore D'Ambrosio Lettieri, riguardante le professioni, che francamente poco concernono il tema di cui trattiamo. Si tratta di temi che sarebbe molto opportuno esaminare nelle Commissioni di merito in provvedimenti che si occupano di queste specifiche materie. Sotto questo profilo il parere del Governo è contrario alla trattazione di ulteriori temi all'interno

di pari tenore rispetto al contenuto del provvedimento.

del testo proposto dalle Commissioni riunite, formeranno oggetto di un autonomo disegno di legge (1082-*bis*), dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

dal titolo «Delega al Governo per il riordino delle funzioni del segretario comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Presidente, insisterei per l'accantonamento

Ciò crea un problema molto grave sull'autosufficienza riguardo alla disponibilità di sangue e di emoderivati, segnalata dal Centro nazionale sangue e condivisa dallo stesso Governo.

francamente trovo inconcepibile che in un decreto sulla semplificazione venga introdotta una norma grazie alla quale viene eliminato il principio di reciprocità nell'ambito delle vendite nel settore degli emoderivati. Si tratta di un principio fondamentale e semplicissimo: le imprese straniere possono vendere in Italia a condizione che le imprese italiane possano vendere nei Paesi da cui provengono le imprese straniere.

Chi parla al telefono, chi discute, chi si muove, chi dà le spalle, c'è di tutto oggi in quest'Aula! Presidente, la questione è diversa. Noi abbiamo lavorato in regime di monopolio fino al 2005. La motivazione per cui fu varata la legge voglio ricordarlo - fu proprio quella di consentire una diversa identificazione delle aziende che operano sul territorio nazionale, ma che trattano il plasma anche al di fuori dei confini italiani, in maniera da assicurare pari opportunità e soprattutto per raggiungere un equilibrio di autosufficienza nel settore degli emoderivati. Chi conosce bene la materia sa che è proprio per questo vincolo

è difficile in questa sede esprimere un parere con chiarezza, tanto più che riguarda un Dicastero diverso da quello che ho l'onore di rappresentare. Giustamente il senatore Tomassini ha detto che sarebbe opportuno esaminare la materia nell'ambito della Commissione sanità, ragionamento che condivido. Mi domando se c'è modo di esaminare l'emendamento in titolo in Commissione compatibilmente con i tempi di questo provvedimento che, malgrado tutto, è pur sempre un collegato e dovrebbe entrare in vigore entro una data plausibile, se non rapida. Quindi, mi permetto di insistere

articolata sulla scelta della tematica degli emoderivati. Sono state formulate anche obiezioni sul principio di reciprocità; è un tema che va discusso e credo che la competente Commissione potrà

e considerata anche la grande attualità di un problema che è nella più alta priorità dell'attenzione non solo politica, ma anche delle organizzazioni del settore,

forma all'ordine del giorno G3.124 che è stato accolto dal Governo, nella persona del sottosegretario Vegas, in sede di L'urgenza - così come avevo già detto in quell'occasione - è dovuta al fatto che numerose imprese che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della legge n. 388 del 2000 si trovano ad affrontare da alcuni mesi gravissimi problemi a seguito appunto della comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria della perdita del beneficio fiscale, già interamente compensato, per mancato invio del modello CVS. Comprendendo quindi la gravità della paralisi finanziaria che si viene a determinare per queste imprese, anche considerando il momento di crisi che sta vivendo il Paese, particolarmente nel Mezzogiorno, in sostanza si dà questa interpretazione autentica limitatamente ai soli soggetti ricompresi

stabilire che il blocco dei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni per importi superiori ai 10.000 euro è sospeso nel caso ci sia il ricorso del beneficiario fino alla sua definizione.

a cui corrisponde la relativa copertura finanziaria, e lasciare soltanto il comma 1, che non fa altro che riprendere alla lettera un ordine del giorno che il Governo ha già approvato in sede di manovra finanziaria.

affronta una problematica reale, peraltro già oggetto di un ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo; pertanto, anche se avere due ordini del giorno sulla stessa

Colleghi, la seduta è ripresa, vi prego di prendere posto.

L'asta elettronica è uno strumento molto importante, che consente alle pubbliche amministrazioni un notevolissimo risparmio. Oggi, le pubbliche amministrazioni che lo usano sono poche, ma quelle poche che lo usano ottengono risparmi notevolissimi.

Soprattutto in questa situazione economica, signor Presidente, e mi rivolgo anche al Governo e al relatore, ciò vuol dire aprire di più il mercato e renderlo accessibile, per

mi riallaccio alla discussione che abbiamo svolto con il relatore e il rappresentante del Governo in relazione al precedente emendamento concernente le imprese artigiane. Qualora vi sia la conferma di un parere favorevole, direi di non dilungarci oltre ma di portare a casa il risultato nell'interesse delle imprese artigiane. che per intese raggiunte tra i colleghi Capigruppo la seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 19.

12.0.5 (testo 2), che non è accoglibile in quanto fa riferimento ad un istituto che non può essere preso come parametro in una valutazione di legge.

Esso regola la possibilità di piccole imprese artigiane, anche in caso fossero consorziate in consorzi stabili, di partecipare alle gare

ci si riferisce ad importi di lavori inferiori a 10 milioni e ad importi di forniture inferiori a 2 milioni. Gli articoli che andiamo a modificare si riferiscono invece a importi di lavori

Signor Presidente, premesso che - ahimè - per quanto riguarda il turismo, si continua a perseguire la strada della disorganicità e si introducono provvedimenti qua e là nei vari decreti e che se si continua così difficilmente si riuscirà a dare ordine alla materia e rilancio ad un settore che langue e rischia di sprofondare,

fossero destinate allo sviluppo del settore del turismo e al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive. Con questo articolo il Governo cambia, dirottando lo stanziamento su non meglio precisati progetti di eccellenza e di competitività.

che intendono sollecitare l'attenzione del Governo su un problema serio. Sono stati operati tagli molto pesanti in finanziaria sulla gestione della navigazione dei laghi. Non trasformo nemmeno questo emendamento in un ordine del giorno, onorevole Vegas Vegas (so che lei porta la croce; è costretto a cantare e a farlo anche in modo intonato, quindi sa che non è una questione personale), perché non c'è il tempo per impegnare il Governo su qualcosa di concreto. E le spiego perché. Questi tagli porteranno nelle prossime settimane ad una forte riduzione delle corse dei dei battelli e quindi del trasporto pubblico lacuale e probabilmente determineranno anche una riduzione del numero dei lavoratori stagionali, pari a 160. La questione è particolarmente delicata. Ringraziamo il ministro Matteoli che si è messo immediatamente a disposizione. Quindi ritiriamo l'emendamento perché con il ministro Matteoli stiamo

che lavorano per nove mesi, dopodiché ritirano il TFR con cui vivono per tre mesi per poi essere nuovamente riassunti. Condividiamo la vostra politica dei tagli, per quanto riguarda i cosiddetti rami secchi. Però le posso garantire, Signor Sottosegretario, che se c'è una gestione virtuosa è proprio quella della navigazione dei laghi. Quindi ringraziamo ancora il ministro Matteoli per l'attenzione che ci ha manifestato e speriamo molto presto di risolvere questo problema.

come bene ha illustrato ieri il senatore Zanda, voglio esprimere preoccupazione per quel che si vuol fare dell'ENIT: prima lo si riforma, poi si nomina un presidente, poi si si riducono pesantemente i fondi a disposizione. Con questo articolo 12-*ter* si riconducono i membri da 13 a 9, e su questo si può essere anche d'accordo; però poi si introduce un concetto di commissariamento, senza peraltro indicare un tempo entro il quale

Queste somme vanno a ridurre gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa, di cui al comma citato.

si pongono l'obiettivo di tenere ferma la volontà del legislatore di ristabilire l'incompatibilità tra iscrizione all'albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, cioè l'articolo 1 della legge 25 novembre le posizioni acquisite *medio tempore*, i cosiddetti diritti acquisiti, tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1,

Tutto ciò è stato comunicato al Ministero della giustizia e a quello dell'economia e delle finanze dal Consiglio nazionale forense in sede di esame di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ma che poi evidentemente non ha concluso il suo *iter*. Quindi, con questo emendamento si supererebbero i seri problemi di incostituzionalità

Sarebbe meglio affrontare il tema nella sede propria e non in questo provvedimento. Quindi, vi è un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno, che sarebbe accolto dal Governo come raccomandazione.

«Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari. Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale

del tutto sottratto al controllo del Parlamento che pure ha istituito per legge tali società, esse sono state invitate a mettere in liquidazione l'INSAR. L'emendamento, se approvato, dispone il passaggio delle quote azionarie alla Regione Sardegna, che è ben lieta (anche nella nuova interpretazione politica nelle mani del nuovo presidente della Regione, eletto due settimane fa)

questa società, alla quale il Parlamento italiano ha conferito delle risorse per fare politiche di intervento sul lavoro nel Mezzogiorno, restituirà i soldi ad altre società, come Fintecna

Il commissario straordinario è stato nominato anche a causa del dissesto finanziario. La Croce Rossa italiana, attraverso le convenzioni, deve recuperare autonomamente i finanziamenti per il personale Si dice che non bisogna ulteriormente caricare sul bilancio dello Stato. Purtroppo, si tratta dell'intero *deficit* della Croce Rossa italiana e siccome questo ente è ancora commissariato, penso che il Governo abbia il tempo di verificarne bene l'organizzazione, la gestione,

far notare tanto al rappresentante del Governo quanto al relatore che abbiamo preso una direzione chiara in questo provvedimento: vogliamo andare incontro all'utente nei confronti delle grandi organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi pubblici essenziali o di pubblica Se prendiamo però la strada del sostegno ad una giustizia rapida e non costosa, cioè la via della conciliazione,

si dà una propria regolazione, questa esce completamente dalla possibilità di adire a vie alternative conciliative; altrimenti tutti i grandi enti che gestiscono servizi pubblici adotteranno

di conciliazione prevedendo la rigidità e il controllo da parte del Governo, nonché la rapidità (si danno al massimo quattro mesi per definire le procedure), questa è una buona cosa che faremmo nei confronti dei cittadini. Non vorremmo perdere questo treno, sarebbe un peccato.

l'importanza di sentire le associazioni dei consumatori proprio in relazione alla tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici. Questo articolo prevede, infatti, per categorie di utenti che lamentino la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione stragiudiziale della controversia. L'emendamento 21.6 andava proprio nel senso di sentire le associazioni dei consumatori nel momento in cui veniva emanato un decreto che individuava uno schema tipo di procedura

la data per le elezioni amministrative ed europee possa comportare un costo di oltre 400 milioni di euro. In un contesto in cui le casse dello Stato piangono miseria,

dovrebbe essere chiaramente spiegato da questo Governo. Volevo quindi ricordare che esiste un'interpellanza firmata da decine di senatori.

vorrei ancora una volta - sinteticamente, ma con grande forza - portare all'attenzione di quest'Aula la grave e drammatica situazione in cui versa la FIAT di Pomigliano d'Arco. L'azienda, che è stata per decenni il simbolo dell'industrializzazione della Campania e di Napoli e ha dato occupazione a migliaia di lavoratori, oggi vede paurosamente vicino il tramonto. Abbiamo sottolineato più volte, sia in quest'Aula, sia attraverso varie interrogazioni, l'urgenza di un intervento del Governo sulla FIAT, affinché sia chiarita la missione industriale per questo stabilimento e siano salvate le migliaia e migliaia (quasi 5.000) di posti di lavoro, tra operai e impiegati. Abbiamo chiesto che ci sia un incontro, un tavolo nazionale, sulla FIAT di Pomigliano d'Arco, anche perché gli ecoincentivi pensati dal Governo per dare una risposta alla crisi dell'auto non hanno riguardato lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Una delegazione dei lavoratori, forse qualcuno di voi lo avrà ha lanciato un grido d'allarme recentemente anche attraverso una trasmissione nazional-popolare qual è il festival di Sanremo ottenendo, vorrei dirlo, più attenzione da parte di Bonolis che non sensibilità da parte della politica su questo argomento. Domani ci sarà una ulteriore manifestazione a Pomigliano La Regione Campania ha chiesto un intervento al Governo, al ministro Scajola e al ministro Sacconi, come abbiamo fatto anche noi ma, Presidente, finora ci è parso che l'indifferenza abbia avuto la meglio sull'attenzione. i giornali di ieri riportano ampiamente che il Direttore generale del Policlinico Umberto I è stato condannato dalla Corte dei conti perché si è auto-aumentato lo stipendio, che risulta più alto di quello altri direttori generali di altre strutture, strutture, di policlinici universitari e di aziende ospedaliere. Io ho presentato un'interrogazione su questo e sollecito la Presidenza affinché si venga a riferire

del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,